del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali Il provvedimento si compone di dieci articoli suddivisi in quattro capi. Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del 2021; in particolare, modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento nelle zone bianche e gialle di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, e in altri locali o spazi anche all'aperto. Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi Covid-19, si stabilisce in linea generale che: nelle zone gialle permangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. Un emendamento, a prima firma del senatore Grassi, ha risolto una questione interpretativa sull'ambito di applicazione con riferimento alla non necessità dei posti preassegnati a sedere. Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Un'ulteriore disposizione consente nelle zone bianche lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di areazione senza ricircolo dell'aria. Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono rispettivamente pari al 50 per il venir meno in zona bianca dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati. L'accesso alle strutture in zona bianca è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde; viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico. In caso di violazione delle regole su capienza e *green pass* si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni a partire dalla seconda violazione. Tra le modifiche introdotte si segnala, per i locali da ballo, l'equiparazione agli impianti di areazione di sistemi di filtrazione a elevata efficienza in grado di ridurre la presenza del virus nell'aria (con l'emendamento 1.8 a firma del senatore Perosino).

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico nelle zone bianche e nelle zone gialle dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, fermo restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, che richiede per i lavoratori pubblici e privati il possesso di un certificato verde Covid-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze. L'emendamento del Governo 3.0.1000 ha stanziato ulteriori risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Con il subemendamento 3.0.1000/1, a firma della senatrice Riccardi, la Commissione ha previsto che per le elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre, al fine di favorire il distanziamento, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate. Nel capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali coordinate da un segretario generale; il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15. L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di *referendum* depositate entro il 31 ottobre 2021. La scelta da parte dei promotori del *referendum* sulla giustizia di non depositare le firme, ma di procedere alla richiesta tramite i consigli regionali ha notevolmente semplificato le operazioni di verifica da parte dell'Ufficio centrale. Con l'emendamento approvato 5.2, a firma del senatore Calderoli, sono state ridotte le risorse umane e finanziarie messe a disposizione, concretizzando il risparmio che si voleva ottenere in questo modo. L'articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato dello scorso anno, introduce l'obbligo di *green pass* per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove. Nel capo III, l'articolo 7 incrementa per il triennio 2021-2023 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo (FNPSA), al fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in Afghanistan. Pirovano, approvato dalla Commissione, intende specificare che tali risorse siano destinate ai richiedenti asilo provenienti da quel Paese e non ad altri fini. L'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima università sono assicurate, a compensazione, due immobili, uno dei quali destinato a divenire la nuova sede della richiamata scuola. L'articolo 9, che introduce il capo IV, reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo è stato interamente sostituito da un emendamento del relatore che rappresenta la sintesi tra le sollecitazioni del Garante della *privacy*, le esigenze del Governo di semplificare la materia della tutela dei dati personali per fini pubblici, al fine di accelerare i meccanismi amministrativi anche in funzione del PNRR, e alcune segnalazioni pervenute dai Gruppi attraverso gli emendamenti. Ho ritenuto preferibile presentare un emendamento interamente sostitutivo, piuttosto che procedere a una serie eccessiva di modifiche puntuali, per evitare il rischio di distorcere il significato complessivo della norma, anche in considerazione della possibilità di subemendare il testo per apportare ulteriori miglioramenti, ciò che in effetti è avvenuto con l'approvazione di diversi subemendamenti. In particolare, la nuova formulazione delle modifiche all'articolo 2-*ter* del decreto legislativo n. 196 del 2003, il codice in materia di protezione dei dati personali, assicura maggiori garanzie con l'ampliamento della base giuridica per trattare dati personali nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, comprendendo anche gli atti amministrativi di portata generale, in modo da limitare la discrezionalità dell'amministrazione. Si tratta, peraltro, di una modifica proposta dal Garante per la *privacy* nel corso della sua audizione in Commissione, anche al fine di allineare la normativa italiana al regolamento europeo. Per quanto riguarda la diffusione delle comunicazioni di dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, è previsto che ne venga data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione, per consentire che intervenga con propri provvedimenti. È poi stata inserita una norma specifica sui dati personali relativi alla salute in ragione della loro particolare rilevanza; infatti, in questo caso, è previsto il parere preventivo del Garante, proprio al fine di accrescere la tutela di queste informazioni sensibili. Per quanto riguarda il *revenge porn*, prendendo spunto dall'audizione del procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, è stato inserito un riferimento anche alle registrazioni audio, oltre alle immagini e ai video, di cui è vietata la diffusione. Inoltre, è stato previsto un onere aggiuntivo per i gestori delle piattaforme digitali, che dovranno conservare copia del materiale oggetto della segnalazione ai fini probatori per l'eventuale esercizio dell'azione penale, che ovviamente richiede tempi più lunghi rispetto all'intervento del Garante, che per sua natura deve essere tempestivo e immediato. Tramite subemendamenti il testo dell'articolo 9 è stato ulteriormente migliorato. Ricordo, quanto alle norme sul *revenge porn*, l'estensione a ogni documento informatico nel loro ambito di applicazione, con il subemendamento 9.100/26, a prima firma della senatrice De Petris; la soppressione della necessità di una violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, con il subemendamento 9.100/30 a prima firma del senatore Perilli; l'estensione da nove a dodici mesi dell'obbligo di conservazione del materiale da parte delle piattaforme destinatarie

In ragione delle nuove rilevanti funzioni attribuite al Garante, un subemendamento presentato da tutti i Gruppi ne ha previsto il potenziamento del ruolo organico, con relativo stanziamento di risorse;

Infine, sono state sospese, fino alla fine del 2023, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con il subemendamento 9.100/64 (testo 2) del senatore Ferrari. È stata poi introdotta, come di prassi, la clausola di salvaguardia per le Regioni a

rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la fase acuta e più impegnativa della pandemia è stata gestita dal Governo Conte II, con scelte difficili e drastiche, a volte impopolari, ma necessarie per arrestare la diffusione del virus e sostenere nel miglior modo possibile le attività economiche gravemente coinvolte e sconvolte dall'emergenza pandemica. Il Governo Draghi ha proseguito su questo percorso e, forte del successo della campagna vaccinale e dell'alto l'indice di adesione ad essa, soprattutto se rapportato a quello di altri Paesi europei, ha potuto iniziare il graduale e progressivo processo di ritorno alla normalità, di ripresa di tutte le attività economiche, di riapertura di servizi e strutture, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione e della dovuta attenzione che ognuno di noi deve avere verso la salute altrui. Riprendere una socialità, un modo di relazionarsi che ci coinvolga in emozioni, da vivere e condividere insieme, con la partecipazione ad eventi, avvenimenti, momenti coinvolgenti di sana condivisione collettiva, è stata la speranza concreta e il pensiero struggente durante i momenti più difficili della pandemia. Vedere l'attuale difficile situazione che vivono altri Paesi europei, costretti a *lockdown* più o meno parziali e a dover far fronte a numeri di contagi e di vittime da Covid-19 nettamente più elevati rispetto a quelli attuali del nostro Paese, conferma che il percorso seguito è quello giusto, al di là delle tante difficoltà che realisticamente lo costellano e delle diverse critiche di parte, fatte spesso per cercare consensi e visibilità o per mera propaganda politica. Certamente errori sono stati commessi, ma d'altronde non sbaglia chi non opera o non ha la responsabilità di decidere. Essi sono stati spesso frutto del difficile coordinamento tra le diverse strutture impegnate nell'emergenza o delle problematiche connesse al rapporto tra la cabina di regia centrale e le diverse realtà regionali e locali. occorre andare avanti, con caparbietà e responsabilità e soprattutto seguire le indicazioni della scienza e di chi ha le competenze scientifiche e i requisiti riconosciuti per fare osservazioni e dare giudizi. Occorre farlo non pedissequamente, ma con le opportune considerazioni, elaborazioni e valutazioni politiche, queste ultime frutto, senza dubbio, del confronto fra le diverse anime che hanno la responsabilità di governare e di programmare le scelte e gli indirizzi migliori per il nostro Paese, per portarlo fuori dall'emergenza sanitaria, sociale ed economica che la pandemia ha provocato. Per fare tutto ciò nel modo migliore, però, occorrono lealtà e franchezza nei rapporti e nel confronto tra le diverse forze politiche, pur riconoscendo le differenze più o meno marcate e le diverse opinioni che ciascuna posizione sicuramente comporta. Nonostante ciò, alcune forze politiche hanno avuto spesso posizioni ondivaghe e atteggiamenti altalenanti, frutto spesso di mero calcolo politico, di propaganda elettorale o di valutazioni derivanti dalla variabilità delle percentuali dei sondaggi. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre mantenuto una linea chiara, ferma, decisa e lineare. Non bisogna strizzare l'occhio - come qualcuno fa un giorno sì e un altro pure - ai no vax o accattivarsi i favori e la benevolenza dei no *green pass*. L'unica cosa importante è la tutela della salute del singolo e della collettività e fare tutto il possibile per salvaguardarla, agendo in tale direzione. Come più volte ha ribadito anche il nostro presidente Conte, la tutela della salute pubblica viene prima di ogni altra cosa. Occorre seguire le direttive scientifiche, stimolare, sensibilizzare, informare, diffondere e allargare il percorso vaccinale. Dare grande impulso al *green pass*, come misura di contenimento della diffusione della pandemia, come possibilità concreta di ritorno alla normalità in tutti gli ambiti della vita della nostra collettività e come mezzo di rispetto della salute del singolo cittadino, delle fragilità e delle persone in difficoltà. pure nella possibilità offerta a chiunque di operare scelte diverse e di avere opinioni differenti, che non devono però - questo è importante - essere imposte mortificando o precludendo agli altri, che rappresentano la maggioranza, momenti di socialità o addirittura rappresentando un pericolo o un rischio per la salute

e che rappresentano la linfa vitale dei provvedimenti presenti nell'agenda politica.

al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, per le ennesime e gravissime minacce, ricevute in modo diretto e palese da terroristi dell'ISIS. Vicinanza e sostegno a Luigi Di Maio che, nel suo delicato ruolo istituzionale, dimostra, con il suo impegno e le sue azioni concrete, che l'Italia è in prima linea contro il terrorismo e non arretra di fronte a questi vili messaggi intimidatori. Le minacce dell'ISIS al nostro titolare della Farnesina confermano ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, il grado di esaltazione mentale, la spregiudicatezza e le deplorevoli azioni aggressive di menti perverse, in preda ad apparenti deliri mistici di esaltazione, ma in realtà assetate di violenza, di odio e di sangue, che trovano radici in un paradiso religioso becero e asservito a false ideologie. La nostra risposta deve essere ferma, decisa e unanime. Il nostro Paese è in prima linea nel processo di stabilizzazione internazionale ed è unito di fronte alla violenza da qualsiasi parte provenga. Siamo tutti con Luigi Di Maio e a difesa della sicurezza del nostro Paese.

l'intervento odierno si è reso necessario per parlare di un decreto adottato nell'ambito della complessa gestione della curva epidemiologica nel nostro Paese. Apprezzo con piacere che, anche su questo tema, il Governo Draghi si è mostrato e continua a mostrarsi in continuità con il Governo Conte. In continuità nel senso che ha proseguito e dato seguito a quanto fatto sin dalle fasi iniziali della pandemia, con la differenza che nel marzo del 2020 andavamo incontro all'ignoto mentre oggi conosciamo meglio il nemico e disponiamo anche di armi più efficaci per combatterlo. Mi preme sottolineare anche altri aspetti di continuità tra Governo Conte e Governo Draghi, nella misura in cui il secondo esiste solo grazie ai traguardi conseguiti dal primo. A tal riguardo, non posso non citare il fondo garantito dal bilancio dell'Unione europea. Al netto delle false motivazioni presentate lo scorso inverno, magicamente sparite dal dibattito politico e dai rulli delle agenzie, appare chiare che l'intento di gran parte dell'emiciclo parlamentare era quello di poter gestire gli oltre 200 miliardi ottenuti da Giuseppe Conte e di potersene prendere i meriti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, colleghi. Mi pare giusto e corretto, nonostante la narrazione interessata tenti di disorientare. Ma tant'è: ribatteremo con caparbietà e tenacia per rivendicare la bontà del nostro lavoro. Ancora, sono già numerosi gli annunci e i proclami da parte di Ministri e Sottosegretari, che non hanno perso tempo ad annunciare la partenza di progetti finanziati proprio grazie ai fondi ottenuti solo per merito della caparbietà di Conte e del MoVimento 5 Stelle e non mi risulta difficile pensare che questa sarà la tendenza, almeno fino alle elezioni del 2023. D'altronde il Governo Draghi, di fatto, si sta occupando del ritorno alla normalità, con i contagi sotto controllo, sebbene in lieve crescita, e dell'attuazione del PNRR e quindi, in sostanza, sta costruendo sulle solide fondamenta poste dal precedente Esecutivo, senza le quali oggi l'Italia non avrebbe questa grande occasione di rilancio. Onorevoli colleghi, neanche il decreto-legge in discussione fa eccezione. D'altronde non è passato molto tempo da quando sono intervenuto in quest'Aula annunciando la necessità, in favore di cittadini e imprese, di procedere senza esitazioni a nuove riaperture, soprattutto una volta terminati gli effetti dei ristori, ed è proprio questo che si prefigge il decreto-legge in esame. Con tale provvedimento, infatti, che introduce nuove disposizioni all'interno del decreto-legge n. 52 del 2021, il cosiddetto decreto riaperture, è stato finalmente possibile procedere alla riapertura al 100 per cento della capienza, sia all'aperto che al chiuso, in zona bianca, di teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di cultura, locali di intrattenimento e musica dal vivo, ma anche di sale da ballo e discoteche, al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso, e siamo anche tornati a riempire palazzetti e stadi. numeri e percentuali che non rendono l'idea di cosa significhi esattamente questo provvedimento. Pensate che in molti casi si tratta di attività rimaste chiuse sin dall'inizio della pandemia: cito, ad esempio, il caso più eclatante, quello delle discoteche e delle sale da ballo, che sono rimaste chiuse per quasi venti mesi, praticamente senza soluzione di continuità. Parliamo di circa 3.000 attività e oltre 100.000 posti di lavoro e dunque non dobbiamo soltanto pensare al fine ludico di chi ne fruisce, ma alle migliaia di famiglie che vivono grazie a queste attività e che per tutto questo tempo sono rimaste prive di lavoro, nonché della loro fonte di reddito. Del tutto inopinatamente, dal decreto-legge era rimasto escluso il settore fieristico e congressuale, l'unico che soggiace ancora ai limiti di capienza del 50 Come MoVimento 5 Stelle abbiamo deciso di dare immediato riscontro alle loro istanze e durante l'esame in Commissione, insieme ai senatori Croatti e Toninelli, pur ritirando l'emendamento 1.15 e i testi successivi, con cui si intendeva portare al 100 per cento la capienza consentita per convegni e congressi in zona bianca, abbiamo ottenuto l'approvazione di un ordine del giorno vincolante - lo ripeto: vincolante - che recepisce tale istanza, che va risolta entro il 30 novembre. Per quanto riguarda le fiere, in questo ordine del giorno approvato si consente il loro svolgimento in presenza anche su aree pubbliche, tanto in zona bianca, quanto in zona gialla, senza restrizioni in termini capienza, purché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. Al fine di consentire la piena partecipazione agli eventi fieristici, viene inoltre garantito il libero ingresso dall'estero nel territorio nazionale, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza. Il provvedimento in esame, però, non può e non deve essere considerato avulso dal concreto andamento della curva epidemiologica e degli altri parametri di allerta in grado di determinare il grado di rischio per ciascuna Regione. Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad una crescita dei contagi, che non va sottovalutata. Bene dunque le riaperture, ma non si abdichi ai controlli, che devono essere ancora maggiori, per garantire il rispetto delle misure precauzionali rimaste a scongiurare in tutti i modi nuove restrizioni. Con l'auspicio, per tutti noi, di non doverci più trovare a discutere di questo genere di decreti e di poter finalmente dedicare la totalità dei nostri lavori alla crescita economica e al rilancio dell'Italia, si continui dunque con la legge di bilancio a trovare soluzioni per i cittadini, senza dimenticare il superbonus, che sta subendo attacchi immeritati. Complicare le cose semplici pare un'attività che va per la maggiore, ma il MoVimento 5 Stelle, con l'aiuto dei portatori di buonsenso, non lo permetterà e si impegnerà a rendere comprensibile una misura che tanto sta facendo per l'efficientamento e il miglioramento delle case degli italiani. Grazie e buon lavoro a tutti noi, con particolare riguardo ai portatori di buonsenso.

alla conversione in legge del decreto-legge n. 139, che è stato chiamato decreto capienze, ma in realtà soltanto un articolo può riferirsi al titolo del provvedimento, che ha modificato, aumentandolo, l'accesso ai luoghi pubblici sia all'aperto, sia al chiuso, per quello che riguarda lo spettacolo, sia esso riconducibile all'intrattenimento, alla cultura o allo sport.

parlare di tanti altri argomenti all'interno di questo provvedimento, che solo casualmente può definirsi decreto capienze. Ci troviamo di fronte a una melassa indistinta di argomenti distinti e distanti tra di loro,

ad affrontare, invece, in maniera frettolosa e nell'indifferenza generale dell'Assemblea, una serie di argomenti che - lo ribadisco - avrebbero meritato un'attenzione diversa. Questa è l'ennesima mortificazione nei confronti del Parlamento, che noi di Fratelli d'Italia vogliamo denunciare con forza. La prima, quindi, è una severa critica di metodo nei confronti di questo provvedimento. Come dicevo, un solo articolo un solo articolo è riferito alle capienze; gli altri hanno iniziato a spaziare dalle problematiche del Ministero della salute per passare agli uffici agli uffici centrali del *referendum*, agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza Covid e, ancora, all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

sollevare alcuni rilievi circa taluni aspetti dell'unico articolo che invece ha ritenuto di affrontare, sotto il profilo dell'emergenza epidemiologica, temi riconducibili alla frequenza di alcuni luoghi pubblici.

sono comunque condizionate - questo ovviamente vale per tutti i contesti della vita pubblica - all'esibizione del *green pass.* fortemente la possibilità di arrivare a ottenere cifre accettabili all'interno dei luoghi che hanno ospitato questo tipo di di manifestazioni, che - salvo rare occasioni - hanno permesso il raggiungimento di un tetto di pubblico sufficiente, perché appunto la limitazione del *green pass* ha inevitabilmente prodotto difficoltà per l'accesso a questi luoghi.

Il provvedimento in esame avrebbe meritato di essere trattato in maniera diversa, se non altro perché alla frequenza degli stadi - e qui mi riferisco allo sport professionistico - sono legati alcuni aspetti collaterali, come dicevo poc'anzi,

dall'attività calcistica su tutto il movimento sportivo nazionale. Questo è accaduto dal dopoguerra ad oggi: addirittura sino al 2000 il mondo del calcio, attraverso il Totocalcio, è riuscito a produrre risorse necessarie per il mantenimento di tutto il mondo dello sport. Dal 2000 in poi, invece, il contributo pubblico è stato agganciato al gettito fiscale prodotto dal mondo del sport, per poi riversare, attraverso contributi, i sostegni necessari al mondo dello sport stesso, fino ad arrivare ai giorni nostri, al 2018, quando la legge di bilancio ha modificato l'ordinamento sportivo nazionale, individuando nel 32 per cento del gettito fiscale prodotto dallo sport

difficoltà sopravvenuta per gli effetti post-pandemici, che hanno generato una crisi finanziaria in tutti i comparti della società civile, in particolare nel mondo dello sport, si aggiunge l'impossibilità di mantenere misure ordinarie che non è stato possibile assicurare attraverso l'afflusso regolare agli stadi e questa misura lo ha confermato. Ci troviamo pertanto di fronte non solo all'impossibilità di riavviare in maniera ordinaria l'attività, ma anche a un provvedimento che di fatto limita

alla legislazione sugli stadi, che è carente e insufficiente, alle agevolazioni fiscali, che non sempre vengono concesse nei confronti delle attività sportive, e al sistema dei diritti televisivi, che è obsoleto e inadeguato rispetto alle esigenze di questo importante settore. Il tutto rende

criteri attraverso i quali si va a reimmettere linfa all'interno dello sport italiano, aumentandola e riportandola alla misura ordinaria del 100 per cento, pur subordinandola al *green pass*.

Ieri il numero dei contagiati in Italia è stato pari a 10.172, con 72 morti, 6.406 guariti, cinque posti occupati in terapia intensiva in tutta Italia e 90 ricoveri. Questi sono i dati sulla base dei quali si stanno comprimendo i diritti costituzionali dei cittadini, tra cui quello

Con il provvedimento oggi in esame si sdogana la possibilità per i funzionari della pubblica amministrazione di accedere ai dati coperti da *privacy*

che sta gestendo questa presunta fase di emergenza (perché, a questo punto, non possiamo parlare con alcuna certezza) in maniera totalmente arbitraria e fuori da ogni dettame della scienza.

che l'acquisizione preventiva di un foglio di carta dove c'è un QR *code* non corrisponde affatto alla sicurezza sanitaria oppure all'immunità del possessore di quel QR *code* che ha consegnato

nonostante la positività del suo detentore, perché sappiamo che il *green pass* non viene nemmeno sospeso a chi si

a quell'emergenza sanitaria in nome della quale si stanno facendo tutti questi atti sconsiderati. Il Governo ci sta dicendo, attraverso l'informazione pubblica,

e passa al 50 per cento o al di sotto, quindi c'è la necessità di fare la terza dose. Ancora non ho visto un provvedimento

anche la possibilità di accertare lo stato vaccinale dei minori, che, per esempio, nelle scuole sono soggetti a

se in una classe ci sono due ammalati di Covid oppure due casi di positività, gli studenti vaccinati con tampone negativo possono continuare a frequentare, mentre quelli non vaccinati, seppure con tampone negativo, devono essere

vorrei delle spiegazioni a queste misure che si stanno votando e che si stanno esibendo in tutte le sedi attraverso circolari e atti

si devono giustamente scudare i dirigenti per tutti gli abusi che compiranno ai danni dei dipendenti e degli studenti, in qualsiasi sede. tal modo tutto il macroscopico circo che si è venuto a creare su questa emergenza, che ormai solamente da una narrazione del Governo trasmessa a reti unificate da tutti i *media*, che ci stanno bombardando anche con informazioni che provengono da altri Paesi, ma noi stiamo lavorando in questo Paese.

Vorrei porre all'attenzione di quest'Assemblea il livello a cui siamo arrivati: abbiamo veramente superato il livello di guardia; stiamo arrivando a una compressione ormai praticamente totale dei diritti costituzionali, in nome di un'insensatezza, di un'illogicità, di un'irrazionalità scientifica e di una narrazione che proprio non stanno in piedi da alcuna parte. Vaccini Vaccini che addirittura non offrono copertura nemmeno con la terza dose - i contagi circolano anche con le terze dosi nelle RSA e nelle strutture sanitarie - non possono essere una buona giustificazione per condurre una campagna di odio e di disinformazione come quella che questo Governo sta tenendo in piedi per attuare misure

voglio iniziare il mio intervento plaudendo all'attività di questo Governo e di questa maggioranza, non foss'altro per il fatto che siamo passati dall'era dei DPCM, dei DPCM, provvedimenti amministrativi che in sostanza tagliavano fuori il Parlamento da qualunque intervento e giudizio di sindacabilità, a quello dei decreti-legge, che, pur essendo di iniziativa governativa, sono sottoposti al vaglio del Parlamento e in più di un'occasione vengono modificati - dal nostro punto di vista, in meglio -

La strada della vaccinazione - per quanto possibile, di massa - si è rivelata efficace: anche se la pandemia non è completamente debellata, credo di poter dire - e i dati ci confortano in questo - che il peggio è alle nostre spalle. Quanti in questi due anni hanno criticato, anche ferocemente - l'ultimo intervento che mi ha preceduto si inserisce in questo solco - il Governo italiano, e quindi la maggioranza che lo ha sostenuto e che lo sostiene,

che i nostri sacrifici non sono stati vani. Se oggi l'Italia è presa ad esempio dal mondo occidentale, evidentemente questo è merito delle attività che si sono predisposte e anche dell'incentivazione alla campagna vaccinale. Certo, fino a quando non sarà completamente debellata la pandemia, dovremo imparare a convivere con il virus, senza sottovalutarlo, ma senza paura, rispettando le minime regole di distanziamento, utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani,

la possibilità di contagio, sicuramente ne elimina gli effetti più gravi. Qualche giorno fa, leggevo su un giornale

c'erano stati 270 decessi, oggi ne abbiamo avuti poco più di 60 o 70. Questo sta a dimostrare che la vaccinazione è efficace: non è esaustiva, ma è efficace. Altri istituti scientifici hanno potuto accertare che, grazie alla campagna di vaccinazione, abbiamo salvato la vita a circa 12.000 connazionali: credo che questo sia un risultato assolutamente importante, che non può essere sottaciuto. Proprio per questo mi sia consentito, con tutto il garbo, ma con tutta la decisione necessaria, di invitare coloro che ancora non si sono vaccinati a farlo e a fidarsi della scienza e delle scelte di questo Governo, che non è un Governo di irresponsabili, e di questa maggioranza, che non è una maggioranza di irresponsabili. E proprio perché rivolgo questo invito a coloro che ancora non hanno fatto il vaccino, a maggior ragione invito coloro che hanno fatto le due dosi a fare tempestivamente la terza, perché questa è la strada che dobbiamo seguire fino a quando non avremo debellato completamente la pandemia. Se oggi, grazie a Dio, non parliamo di *lockdown*, fenomeno che invece sta interessando altri Paesi vicini e che stato una fase che ci ha profondamente feriti, lo dobbiamo alle scelte coraggiose di questo Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene, e anche - dobbiamo dirlo - al senso di responsabilità degli italiani. oggi l'Italia è un esempio da imitare e di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi, Parlamento, Governo e italiani, poiché è un risultato di tutti, quindi ne dobbiamo andare assolutamente orgogliosi e fieri. Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire non è soltanto la logica conseguenza dei sacrifici che abbiamo fatto, ma è l'adesione del Governo alle istanze di quanti, Forza Italia *in primis*, chiedevano un ritorno alla normalità, sebbene con tutte le cautele del caso. Teatri, cinema, concerti e musei tornano ad essere attività normali per gli italiani: gustare una partita in presenza o una manifestazione teatrale e vedere un film

Abbiamo un aumento dei contagi e già si parla di ulteriori iniziative e restrizioni che si possono rendere necessarie. Siamo d'accordo che questa dev'essere la strada da perseguire, ma su una cosa vogliamo essere chiari: eventuali responsabilità e restrizioni non potranno mai riguardare coloro che si sono vaccinati, su questo vogliamo essere assolutamente chiari! Abbiamo lasciato libertà e libero arbitro, ma chi ha deciso per motivazioni sue (rispettabilissime, anche se non condivisibili) di non vaccinarsi non può caricare l'onere e le responsabilità di questa scelta su quanti invece responsabilmente hanno deciso di farlo. Questo dev'essere invece un motivo per il quale chi ancora non ha raggiunto il convincimento di vaccinarsi

La presidente Bernini ha commentato in questa maniera: grande soddisfazione per il decreto-legge del Governo sulle riaperture, che ha il marchio di Forza Italia, perché calibra la necessaria prudenza anti-Covid con le sacrosante istanze delle categorie più penalizzate. Non è questa la dichiarazione di voto che, da par suo, farà il collega Pagano, ma credo che si capisca quale sarà l'atteggiamento di Forza Italia di fronte alla conversione del decreto-legge

stiamo convertendo l'ennesimo decreto-legge e siamo reduci dall'ennesima votazione di fiducia: indubbiamente l'attività del Parlamento è ormai ridotta ad un ruolo frammentario e inevitabilmente diventa difficile affrontare in modo organico la trattazione di questi provvedimenti. Proprio in ragione di tale difficoltà, in

Sono ben consapevole - questa è la mia prima legislatura - di essere tornato studente, perché la politica è un altro mestiere rispetto a ciò che possiamo fare prima di questo lavoro, però però non sono immemore delle mie radici e delle mie esperienze. Ho destinato la mia vita alla formazione dei giovani, che continuano ad essere la mia principale preoccupazione. Per il lavoro che svolgo al di fuori di quest'Aula, ho avuto l'onore di partecipare a svariate commissioni concorsuali: ho partecipato a due commissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense, ad alcune commissioni per concorsi universitari e, da commissario, al concorso per uditore giudiziario, cioè per la magistratura. La nostra Carta costituzionale ricorda che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma in realtà - se guardiamo bene - è fondata sull'iniziativa privata - che, vivaddio, c'è e sostiene questo Paese - e anche sui pubblici concorsi, pubblici concorsi, che, a mio giudizio, sono un problema per i giovani e per questo Paese. Parlo per esperienza diretta. I pubblici concorsi soffrono di mancanza di trasparenza. I candidati spesso vengono esclusi senza capirne le ragioni e le commissioni rimangono l'arbitro assoluto

Sappiamo, in ordine a questo decreto-legge, che l'esame di abilitazione alla professione forense è stato conformato

in pratica, al candidato la commissione somministra dei quesiti, ossia questioni concrete da risolvere, a cui il candidato deve rispondere

come le commissioni, al di là dei criteri generali buoni per tutti gli usi, non dovessero rendere pubblici i criteri concreti di valutazione, cioè come a loro giudizio andassero svolte Ho allora tentato in questa sede di introdurre un principio. Ho proposto un emendamento secondo il quale, formulati i quesiti, alla fine della procedura di valutazione la commissione deve pubblicare le risposte, ancorché in modo sintetico. Qual è - o, meglio, qual era - lo scopo di questo emendamento? Imporre alle commissioni rigore, perché tutti coloro i quali hanno partecipato a questa prova sanno che il suo esito è fortemente disomogeneo non solo da Regione a Regione, ma addirittura all'interno della stessa corte d'appello d'appello e della stessa commissione, che - come noto - si articola in moltissime sottocommissioni. Ed è noto che, a parità di svolgimento della prova, qualcuno viene promosso e qualcuno viene bocciato. Perché è un danno per il Paese tutto ciò? Qualcuno potrebbe dire che, alla fine, quello che conta è che si faccia una selezione. È un danno, perché diamo ai giovani la sensazione - anzi, la certezza che le regole lì fuori, quelle che loro devono affrontare usciti dall'università, sono liquide, fluide e mutevoli e passano anche il principio e l'idea che, in fondo, ci si debba far raccomandare, altrimenti quel mondo là fuori diventa una giungla.

in che modo andasse risolto il quesito, per esempio, sul contratto preliminare o quale fosse la risposta corretta a una domanda in tema di usucapione; se facciamo passare questo principio, innanzitutto vincoliamo le commissioni al rigore e alla serietà e facciamo passare il messaggio che questo Paese dà ai ragazzi e ai giovani

ma è chiara la preoccupazione: non introdurre un precedente. Una volta un commissario concorsuale, appartenente ad altro ordine professionale, di fronte a queste mie osservazioni sulla necessità di motivare le bocciature, mi disse: disse: se motiviamo, poi impugnano. Non è un argomento, non è una valida ragione. *(Applausi)*. Sulla base di questo principio la pubblica amministrazione non dovrebbe mai motivare i suoi provvedimenti e i giudici non dovrebbero mai motivare le sentenze. Ma vi dirò di più. Qualche concorso pubblico che impone alla commissione di motivare c'è ed è anche un concorso estremamente selettivo, che regala a questo Paese una classe professionale di grandi capacità: è il concorso notarile, che è uno dei tre grandi concorsi che si possono affrontare dopo la laurea in giurisprudenza. La commissione del concorso notarile deve motivare le ragioni della bocciatura. Eppure, il notariato, ciò malgrado, da anni serve in modo egregio questo Paese. Quindi, non si deve aver paura di introdurre, come criterio generale, quello della massima trasparenza dell'operato delle commissioni. Noi, in generale, possiamo riscrivere le regole dei concorsi; possiamo prevedere - ad esempio - in ambito universitario, che le commissioni siano frutto di sorteggio o siano composte da personale straniero. L'unica vera arma che abbiamo per far sì che i concorsi siano giusti è rendere trasparenti i criteri di valutazione, qualunque essi siano. Se non introduciamo una massima trasparenza all'interno dei nostri concorsi, se non rendiamo i lavori delle commissioni delle case di vetro, noi faremo sempre un pessimo servizio ai nostri giovani. Non dimentichiamoci che il futuro del Paese sta nelle mani dei giovani. Noi tutti siamo stati giovani e oggi siamo qua; tra venti, trent'anni in questa Aula siederanno coloro che oggi sono ragazzi. Se sbagliamo nella formazione, falliamo nel nostro compito.

il 9 marzo 2020 il *premier* Giuseppe Conte ha annunciato al Paese il *lockdown*: è una data che avrebbe segnato la storia di questo Paese. Sono passati venti mesi, ma adesso l'Italia naviga su una rotta sicura e ben precisa tracciata dall'allora Presidente. In quel frangente eravamo soli e primi, addirittura nel mondo, a cercare le coordinate di una rotta per portare l'Italia fuori da quella situazione. Contro tutto e contro tutti abbiamo intrapreso quelle che oggi sono linee guida per tutto il Paese, che mettono in sicurezza tutti quanti: la suddivisione in aree colorate, l'uso di protocolli in quasi tutte le attività commerciali, i distanziamenti, l'utilizzo di dispositivi come mascherine e protezioni come l'igienizzazione delle mani o l'uso dei guanti, fermare gli abbracci. È stato veramente difficile in questo Paese intervenire con azioni del genere, ma è stato fatto per preservare i più deboli: un patto fra generazioni - come dice sempre la mia collega Barbara Guidolin - fra giovani e anziani.

in riferimento ai dati della pandemia. Dicevo: contro tutto e contro tutti, e un anno fa nei *talk show* politici e opinionisti attaccavano tutte le manovre che portavamo avanti.

Ora su questa rotta si muove il Governo Draghi; una rotta che con orgoglio abbiamo tracciato noi. Tutti in quest'Aula lavoriamo su questi schemi, su quello che è stato dettato dal lavoro del presidente Conte. Stiamo parlando di riaperture: cento per cento di capienza all'aperto e al chiuso nelle zone bianche. Parliamo di posti vitali per il nostro Paese, come teatri, sale di concerto, cinema, luoghi di cultura, locali di intrattenimento, musica dal vivo, per cento al chiuso e il 75 per cento all'aperto di discoteche. Un passo alla volta stiamo intraprendendo il percorso della normalità, ma con intelligenza. Siamo tornati a riempire palazzetti e stadi. Qualche domenica fa sono andato con mio figlio allo stadio. Ho visto persone diligenti entrare mostrando il *green pass* in file ordinate. Tutte le strutture stanno funzionando in una maniera ottimale grazie a questo procedimento.

Il turismo sposta persone, sposta emozioni. È stato veramente difficile. Non era prevedibile e gestibile un tale percorso. Solo regole certe e organizzazione hanno fatto in modo che questo settore potesse ripartire. Le riaperture graduali e l'attenzione sulle capienze hanno

più di 3.000 aziende, di cui un terzo non riaprirà più; 100.000 lavoratori fermi per più di un anno e mezzo. Gli imprenditori che sono rimasti in piedi, con la schiena dritta,

Grazie al presidente Girotto, abbiamo incardinato un affare assegnato in Commissione per trattare il tema delle capienze quando passerà la pandemia. Usciti da questa situazione, dobbiamo cercare di rilanciare in maniera positiva quel mondo,

Abbiamo presentato un emendamento al riguardo, che il Governo ha trasformato in ordine del giorno vincolante entro il 30 novembre. Speriamo che tale sia, ma lo terremo molto monitorato; un emendamento che consentirebbe lo svolgimento in presenza, anche su aree pubbliche, tanto in zona bianca quanto in zona gialla, senza restrizioni in termini di capienza, purché nel rispetto dei controlli e delle linee guida. Ciò consentirebbe la piena partecipazione ad eventi fieristici. Si garantisce il libero ingresso dall'esterno nel territorio nazionale, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza. Ci fa piacere che il Governo abbia intrapreso questo percorso.

È in gioco l'economia del nostro Paese. Sono in gioco i nostri affetti più cari e le persone più deboli. Un ultimo appello: non disperdiamo tutti i sacrifici che abbiamo fatto negli ultimi venti mesi. Non azzardiamo sul nostro Paese, sulla sua economia, sugli imprenditori e sui commercianti. Non scommettiamo sulla vita dei nostri cari.

*in primis* agli Uffici della Commissione, che sono stati di fondamentale supporto per il nostro lavoro in questi giorni. Vorrei poi ringraziare il sottosegretario, Caterina Bini, per il grande supporto e la pazienza nel seguire

Sileri, il presidente Parrini e tutti i membri della 1a Commissione e in particolare i Capigruppo, che hanno collaborato al buon esito

per cercare di individuare la miglior formulazione e dare piena soddisfazione alle variegate

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.9, 1.17, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.12, 3.1, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Il testo in questione - per chiarezza - recita così: «In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati».

di richiamare solo l'elenco dei luoghi menzionati all'inizio del comma, e cioè di indicare soltanto le sale teatrali, le sale da concerto e così via. Tuttavia, la nostra preoccupazione era che in sede applicativa potesse passare un'interpretazione restrittiva, collegando all'elenco delle sale anche la condizione che gli spettacoli si svolgessero esclusivamente con posti a sedere preassegnati. Questo in virtù del generico rinvio operato dal riferimento

In altri termini, grazie all'emendamento, il testo, laddove menziona le zone bianche, recita così: «In zona bianca, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti (...)». Abbiamo quindi escluso in radice che qualcuno potesse cedere alla tentazione di operare una lettura restrittiva del testo. Lo dico affinché sia chiaro che quello che abbiamo ottenuto non è soltanto un miglioramento stilistico, per una maggiore leggibilità della norma, ma è anche un miglioramento di contenuto, giacché adesso la norma non consente più interpretazioni restrittive da parte di chi, maliziosamente, volesse farlo.

non vorrei creare un problema di ordine sanitario, pur sostenendo la causa del settore dei bus turistici che ha patito un grande difficoltà durante questi due anni di epidemia.

desunto da un emendamento che lei ha ritirato; diversamente, essendo identico a quelli che verranno posti in votazione, verrebbe preclusa la votazione del suo.

i soggetti devono essere muniti delle certificazioni verdi Covid, quindi del *green pass,* altrimenti non si può salire a bordo.

pertanto il vincolo della capienza inferiore non ha più senso. Noi abbiamo dato un'impostazione che mi sembrava patrimonio di tutto il Parlamento, perché su questo argomento non ci siamo mai divisi, siamo sempre stati tutti insieme nel rispetto della salute e dell'assetto economico di questo importante settore. tornare a riflettere sulle motivazioni che oggi portano legittimamente - ci mancherebbe - qualcuno ad averci ripensato. Noi speriamo che non ci ripensino, che questo provvedimento venga approvato e che sia un fatto di giustizia, perché ci sono altre attività molto più a rischio che oggi non hanno nessun tipo di limitazione. I bus oggi sono come una sorta di imbuto: chi sale a bordo ha il *green pass,* chi sale a bordo è garantito dal ricambio dell'aria, chi sale a bordo è garantito da una vigilanza seria e concreta da parte del conducente (e in molti casi sono anche in due, se parliamo dei bus turistici, per le grandi distanze). l'aspetto sanitario sui bus turistici si ha una garanzia: se andiamo lì stiamo tranquilli di non ammalarci; invece, se andiamo da altre parti, probabilmente ancora oggi non abbiamo questo tipo di garanzia. mantengano gli impegni che ci siamo assunti tutti insieme in questo anno e mezzo di grande lavoro sul recupero del valore del sistema turistico italiano,

attualmente, la maggior parte dei pediatri di base per riammettere i bambini a scuola richiede l'esecuzione e e la presentazione di un tampone. Ovviamente questo comporta una frequenza elevata di tamponi, perché esiste una patologia respiratoria non Covid, che è sempre esistita,

Signor Presidente, vorrei che fosse fatta una verifica sul voto precedente, in quanto ancora una volta dobbiamo verificare che alcuni colleghi della zona di Forza Italia continuano a votare per i colleghi

consente di scegliere fra coloro che hanno già maturato esperienza in questo particolare periodo e non obbliga ovviamente a una proroga degli incarichi; semplicemente prevede che le persone che abbiano compiuto

Invitiamo il Governo ad una riflessione suppletiva, perché onestamente non capiamo quali siano le problematiche sanitarie avverse che impongono al Governo di esprimere un parere contrario. Non ci sono oneri per la finanza pubblica, il testo prevede una possibilità e non un obbligo e serve in via transitoria, in un momento di pandemia, a ottemperare a una situazione di emergenza; onestamente è irragionevole, oltre che irrazionale,

confermiamo il sostegno del nostro Gruppo all'emendamento 4.0.1 (testo 2), già sottoscritto da parte dei colleghi Saponara, Rivolta, Pizzol e Lunesu. È oggettivo quanto ha appena dichiarato il senatore Cucca: non c'è aggravio di costi, ma una visione che tiene conto della situazione di emergenza, quando aumenta e quando diminuisce, e, soprattutto, dell'apporto importante al sistema sanitario.

a dare una mano ai bus turistici, ma c'è una responsabilità di forze di Governo che devono seguire una linea. *(Applausi)*. A me fa molto piacere che il Parlamento si prenda questa libertà.

ma non mettono in difficoltà il presidente Draghi, votando come Lega, Forza Italia e Italia dei Vivi o Forza i Vivi, come si chiamano, mettendo così in difficoltà la maggioranza. Questo deve essere messo in chiaro e deve restare agli atti. Quindi, chiedo al Ministro per i rapporti col Parlamento che venga immediatamente avvisato il Presidente del Consiglio di questi comportamenti di alcune forze di maggioranza.

Senatore Castelli, le valutazioni di merito politico non spettano a me. Ricordo a tutti l'articolo 68 della Costituzione, per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

più che attinente. Innanzitutto, vorrei stigmatizzare ciò che è accaduto in Aula e che lei giustamente ha riportato sotto un profilo squisitamente giuridico, cioè che esista un problema all'interno di questa maggioranza e che quel problema si chiami democrazia. Non è un caso, infatti, che sull'unico provvedimento dove non viene posta la fiducia si evidenzino le crepe di questa maggioranza. La seconda constatazione è che non può non può passare il messaggio che chi ha votato contro l'emendamento sui bus turistici oggi sia a favore dell'emendamento sui bus turistici. È nell'evidenza dei fatti che esiste chi perora la causa dei bus turistici e chi, invece, con il

Colleghi! Avete preso troppi caffè questa mattina?

Presidente, c'è un brusio insopportabile in Aula e non si capisce quello che sta dicendo. Consiglio una sospensione dei lavori dell'Assemblea almeno di un'ora, in modo da consentire alla maggioranza di ritrovare l'unità di intenti. a titolo collaborativo, perché in tre votazioni la maggioranza è andata sotto, c'è una confusione insopportabile, la maggioranza litiga tra i banchi e non è possibile lavorare in questo modo. Quindi, vorremmo poter votare in coscienza,

Chi è a favore della proposta di sospensione voterà sì, chi è contrario voterà no. Procederemo con il sistema elettronico, senza registrazione dei nomi.

Colleghi, non si può chiedere il silenzio e poi fare rumore. Ascoltiamo il senatore Casini. Presidente, scusi, mi limito ad una considerazione di buonsenso: poiché c'è stata da parte di una collega Capogruppo del MoVimento 5 Stelle la proposta di una sospensione, prima che questa venisse posta in votazione volevo chiedere una precisazione, perché un conto è - anche per un fatto di cortesia che una Capogruppo chieda una sospensione, che secondo me non si nega mai, limitata nel tempo *(Applausi)*, un conto è se la sospensione significa che la seduta non si fa più e che rinviamo a un altro momento.

e una di una sospensione per la durata di una riunione di Gruppo. Pongo quindi ai voti prima la volontà dell'Assemblea su una sospensione e poi sulla durata della stessa. Essendoci stato un equivalente Capogruppo che invece ha manifestato la sua contrarietà, la dovevo mettere ai voti e così l'Assemblea ha deciso. Invito il relatore

Presidente, il decreto che ci apprestiamo a convertire oggi è un provvedimento che non rivede solo il tema delle capienze nei diversi luoghi, ma tocca in modo trasversale anche la riorganizzazione del Ministero della salute, il temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2021, oltre a prevedere alcune disposizioni urgenti in materia di accoglienza e integrazione nell'ambito della protezione dei dati personali. Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, poiché si preannunciava da tempo un altro passo in avanti verso la normalità, con ulteriori allenamenti delle precedenti misure restrittive imposte proprio per il contenimento del contagio.

Grazie Questo decreto prevede novità rilevanti, come il ritorno fino al 100 per cento della capienza in zona bianca per i concerti, i teatri i cinema, la soppressione dell'obbligo di distanziamento sociale nei musei o l'aumento degli ingressi consentiti negli stadi e nelle discoteche. In sostanza, sono misure che permettono a diversi settori di ripartire davvero. Nei minuti che mi sono concessi vorrei soffermarmi soprattutto sulle previsioni in tema di accesso alle attività culturali, sportive e creative, non solo in qualità di Capogruppo presso la Commissione istruzione, ma anche come responsabile del settore sport del Gruppo cui appartengo. Come Italia Viva-PSI abbiamo a lungo insistito per mesi affinché venissero finalmente rivisti gli stringenti limiti delle capienze. Sono convinta si possa fare ancora di più rispetto a quanto previsto da questo decreto, soprattutto se si intensifica la campagna vaccinale e si procede con l'estensione del *green pass* in tutti i luoghi, come già fatto in queste settimane. Con il *green pass* abbiamo noi per primi maggiori sicurezze, perché sappiamo che le persone che ci stanno attorno sono vaccinate, hanno fatto un tampone o sono guarite dal Covid, ma costituisce anche una maggiore garanzia nei confronti degli altri, senza contare il fatto che il *green pass* è stato e continua ad essere l'unica modalità con la quale ripartire a livello economico e sociale e dovremmo fare davvero fronte comune per estenderne la portata e non per ridurla. Grazie allo straordinario lavoro fatto dal Governo Draghi e, in particolare, al piano vaccinale gestito dal generale Figliuolo, siamo stati in grado di fronteggiare il virus e metterci al riparo da nuove chiusure. Stiamo proseguendo in maniera celere con la campagna vaccinale, proprio partendo dai soggetti più fragili e dal personale sanitario. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità nei confronti di tutti

per l'assunzione di un impegno serio e concreto, finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza per procedere a un ampliamento delle capienze anche per altri luoghi. dobbiamo assumerci questo impegno, perché ci sono settori dell'economia che non si sono ancora ripresi dalla crisi pandemica. Penso soprattutto al settore degli sport *indoor:* la capienza degli impianti sportivi al chiuso deve essere equiparata a quella di cinema, teatri e sale da concerto. Oggi, grazie alla grande corsa della campagna vaccinale e all'estensione del *green pass,* non si possono più fare distinzioni. Cultura e sport, come gli altri settori che sono stati penalizzati dalle chiusure, devono poter riprendere a pieno regime. Gli sport *indoor* sono al collasso; le perdite per incassi mancati e gli introiti degli *sponsor* sono da capogiro. Bisogna riaprire tutto e subito; ne va della sopravvivenza di campionati importanti di alto livello, così come di quelli dilettantistici. Per questo, abbiamo convintamente presentato degli emendamenti finalizzati a innalzare i limiti delle capienze anche nelle zone gialle ed estendere ancora di più il *green pass* come unico strumento che abbiamo oggi per tornare alla normalità. Si badi bene: siamo ben consci, purtroppo, della quotidiana crescita dei contagi e comprendiamo, quindi, la prudenza che ispira anche le parole della sottosegretaria Vezzali, secondo cui è ancora presto per parlare di una capienza al 100 per cento per il pubblico negli impianti sportivi, anche a fronte della conferma arrivata dal CTS. Crediamo però anche che dobbiamo pensare veramente a quello che sta succedendo. Pensiamo alla capienza nel Pala Alpitour di Torino, dove sono in corso le ATP Finals di tennis. Il CTS ha respinto la richiesta di una deroga presentata dagli organizzatori per aumentare del 7 per cento la possibilità di accogliere il pubblico nel palazzetto che ospita questo evento, l'attuale situazione pandemica non lo consente. Dobbiamo però parlare chiaramente. Il settore dello sport, soprattutto quello al chiuso, continua a incontrare forti difficoltà che non sono affrontabili solo con i ristori contenuti nei provvedimenti approvati nei mesi scorsi. Inoltre, la piena capienza degli impianti significherebbe molto, consentendo anzitutto di rivivere dal vivo le emozioni che solo lo sport sa trasmettere. Credo che si colga anche da qui il senso del provvedimento. È stata fatta una scelta da parte del Governo, che Italia Viva-PSI sostiene convintamente, ossia consentire un ritorno alle libertà attraverso lo strumento del *green pass*, almeno fintantoché perduri lo stato di emergenza. Su questo non possiamo e non dobbiamo avere dubbi come maggioranza

che ci permette di tornare nuovamente a lavorare in sicurezza, portare serenamente i nostri figli a scuola e goderci serenamente i momenti di svago che ci vengono concessi dalla musica, dalla cultura e dallo sport. Esprimendo il voto favorevole di Italia Viva-PSI al provvedimento in esame, colgo l'occasione per chiedere un gesto di responsabilità da parte di tutti. Mi rivolgo, dunque, a quei Gruppi che probabilmente, mossi dalla volontà di accattivarsi parte del consenso elettorale, ostacolano lo strumento del *green pass* (lo abbiamo visto nei giorni scorsi anche in concomitanza con l'approvazione del che ha previsto l'esenzione della certificazione verde nei luoghi di lavoro). In un contesto in cui contagi stanno aumentando quotidianamente non possiamo avere dubbi su come procedere. I dati confermano l'aumento dei ricoveri e dei contagi, soprattutto in forma grave, e questo è il frutto di scelte irresponsabili da parte di coloro che potendolo fare hanno deciso di non vaccinarsi, mettendo così in pericolo non solo la loro salute, ma soprattutto quella di chi gli sta vicino. Presidente, dobbiamo evitare che queste scelte possano mettere nuovamente in ginocchio il Paese, costringendo il Governo

concetto che è stato ripetuto più volte nei giorni scorsi dal nostro presidente Matteo Renzi: se si dovesse arrivare a delle restrizioni e a dei *lockdown* anche locali, questi dovranno essere solo ed esclusivamente per i non vaccinati. Non sarebbe giusto penalizzare l'intero Paese. Dichiaro il voto favorevole

ma l'ha detto anche il Presidente della Repubblica con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato, che è il modo con cui la Costituzione prevede che il Presidente possa interloquire con il Parlamento, ricordando sia il dettato costituzionale direttamente, sia le sentenze della Corte costituzionale che impongono che il contenuto di un decreto-legge sia omogeneo.

L'adeguamento prevede un incremento della capienza che viene consentita a seguito dell'emergenza Covid. Questa parte, tra l'altro, nel suo spirito di riapertura finalmente, la condividiamo.

altro articolo a tutela della minoranza slovena, che può essere condivisibile, ma non ha nulla a che fare con i centri di accoglienza, che evidentemente non sono per la minoranza slovena, né tantomeno con la parte del provvedimento che riguarda le capienze degli impianti.

grazie a tutti contro quanto è stato ribadito - perché era già cosa ben nota - dal Presidente della Repubblica nel modo più solenne, e cioè con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato. Quanto al contenuto, ebbene, abbiamo assistito a quello che deve fare il Senato, e il Parlamento in generale,

il centrodestra unito, nonostante le differenze - sappiamo bene che Fratelli d'Italia sta all'opposizione mentre gli altri soggetti politici sostengono il Governo - potendo votare finalmente nella sostanza, sono state migliorate alcune misure. Si è finalmente fatta giustizia sui bus turistici, che hanno la possibilità di avere la capienza che hanno gli altri autobus, peraltro fornendo maggiori garanzie. Il testo su cui il Governo si era intestardito prevedeva, invece, una ingiustificata ingiustificata disparità di trattamento. Siamo intervenuti su un articolo - tra quelli che nulla hanno a che fare con il resto del provvedimento - che, per come era scritto, poteva essere condivisibile, ma giustamente è stato trovato un punto debole. Mi riferisco all'articolo che prevede un ampliamento di 3.000 posti del sistema di accoglienza in ragione dell'emergenza dei profughi dell'Afghanistan. Abbiamo più volte esortato il Governo a fare il possibile non per fare un'accoglienza generalizzata di tutti gli afghani che vogliono andarsene dal proprio Paese, ma certamente per coloro che sono personalmente e specificamente perseguitati, coloro che hanno collaborato con la missione militare italiana in quel Paese asiatico. Ebbene, l'emendamento precisava che quei 3.000 posti in più fossero riservati ai profughi afgani; sembrava una precisazione che dovesse essere accolta da tutti, mentre, sorprendentemente, la parte sinistra della maggioranza di Governo

Vengo al contenuto più generale del provvedimento. La prima parte, sia pure con un adeguamento sotto alcuni aspetti - permangono, tuttavia, disparità spesso ingiustificate, che solo in parte sono state corrette - ribadisce l'uso del *green pass*, soggetto, come tutte le norme che riguardano l'emergenza Covid, a continui andirivieni e modificazioni: si sale, si scende, ci si sposta, si modifica la norma.

certezza delle norme almeno per due-tre settimane, possibilmente per uno o due mesi. Se il Governo è sicuro delle norme che ha imposto e della loro efficacia - e dovrebbe esserne sicuro,

suo intervento presso l'Organizzazione mondiale della sanità affinché questa nascondesse una pubblicazione dalla quale emergevano le sue

se l'Italia avesse avuto un piano pandemico degno di tal nome e se fosse stato messo in atto per tempo, anziché vietare le autopsie e fare una serie di altre cose inspiegabili che hanno avuto degli effetti molto gravi.

del trattamento dei dati personali. Ebbene, oggi il trattamento dei dati personali può avvenire in base a disposizioni di legge e da parte di un certo numero limitato di pubbliche amministrazioni. Con queste modifiche non ci saranno praticamente più limiti a tutte le pubbliche amministrazioni - addirittura vengono inclusi gestori di servizi pubblici locali - che potranno quindi accedere e trattare i dati personali delle persone, senza che queste ne vengano informate (se non dalla pubblicazione di questa legge), in base alla determinazione di tali gestori che il trattamento dei dati personali, cioè mettere le mani sui dati personali anche sanitari di ciascuno di noi, possa essere utile a esercitare le funzioni che vengono loro assegnate. che, proprio in questi tempi in cui la tecnologia entra pesantemente nella vita di ciascuno, sia importante tutelare la privatezza e la riservatezza dei dati personali, come tutti i diritti dei cittadini. La tecnologia va usata per il bene dei cittadini e non per controllarli secondo il concetto di uno Stato occhiuto, padrone dei dei cittadini e che vuole tenerli sotto controllo in ogni momento. Noi siamo perché i cittadini siano tutelati nella loro libertà nell'ambito di regole che vanno rispettate da tutti. Signor Presidente, colleghi e colleghe, è davvero difficile intervenire questa mattina. Avevo già preparato una bozza di intervento ieri mattina, i dati che ci hanno raggiunto in serata mi avevano imposto di cambiare la linea del mio intervento. Ma, signor Presidente, colleghi e colleghe, non posso far finta che non sia accaduto niente in Aula questa mattina;

preoccupante, ma che comunque ci deve far riflettere. Questa mattina è accaduto che su alcuni emendamenti (certamente lei ha fatto riferimento a un articolo della nostra Costituzione che tutti noi rispettiamo e nel quale crediamo),

mettere in sicurezza il nostro Paese. Applaudo sicuramente alla collega Sbrollini, che nel suo intervento dichiara che il suo Gruppo sostiene lealmente e convintamente questo Governo, ma ricordo alla senatrice Sbrollini che per tre volte questa mattina ha votato contro il parere del Governo.

la responsabilità a cui tutti siamo chiamati e che tutti noi continuiamo a richiamare; dov'è andata a finire nel giorno in cui raggiungiamo un'impennata di contagi per Covid nel nostro Paese?

Abbiamo un Paese che soffre da due anni dal punto di vista sanitario, come sappiamo bene, e dal punto di vista economico; abbiamo finalmente un Paese che è sicuramente esempio in tutta Europa (ma vorrei dire nel mondo) per come è riuscito ad affrontare la pandemia. necessario fare un esercizio di memoria, colleghi e colleghe, perché in quest'Aula abbiamo pianto, ci siamo rammaricati, ci siamo disperati, abbiamo invocato il maggiore aiuto possibile per quello che accade da due anni

scorso in questi giorni avevamo molti casi e una grande preoccupazione e il Governo, insieme a tanti di noi, diceva chiaramente che ci attendevano mesi bui e

L'anno scorso parlavamo di questo; quest'anno invece, grazie al Governo che spero sosteniamo ancora tutti, a parte Fratelli Italia che è sempre stato coerente,

anche situazioni facili da cavalcare per avere una percentuale elettorale in più nei sondaggi; non lo abbiamo mai fatto perché per noi quello che paga è sempre stato il rigore, la prudenza e la gradualità. Abbiamo sempre detto di aprire un po' alla volta per non richiudere più, grazie anche al grande impegno nella campagna vaccinale e all'uso del *green pass,*

ancora una volta viene prima la lealtà al patto che è stato fatto con i cittadini, perché la loro sicurezza e il loro interesse deve essere sempre messo prima di qualsiasi bandierina elettorale, di qualsiasi strumentalizzazione. strumentalizzazione. In questo senso, in questi due anni il Partito Democratico ha sostenuto convintamente i Governi che si sono succeduti. Non faccio finta che non ce ne sia stato prima un altro, che abbiamo sostenuto convintamente in un periodo molto difficile. molto difficile. Altrettanto convintamente, con grandissima lealtà, sosteniamo il Governo Draghi e tutto il suo Esecutivo, che - è inutile dirlo - ha messo in sicurezza questo Paese.

Continueremo ad usare la stessa responsabilità, la stessa coerenza e soprattutto la stessa conseguenzialità, perché credo che dobbiamo imparare anche ad essere conseguenti a quello che diciamo, tenendo una linea ferma, non strizzando l'occhio a chi cambia idea ogni giorno. C'è infatti chi vorrebbe un giorno aprire, un giorno chiudere, un giorno aprire a metà o chiudere a metà, a seconda di quello che torna meglio. Per noi la linea è chiara: il Paese che è sicuro dal punto di vista sanitario è un Paese che può recuperare anche dal punto di vista economico. Questo lo dimostrano i dati della sicurezza sanitaria che stiamo raggiungendo, che dicono che possiamo riaprire i cinema, i cinema, i teatri e gli stadi. Torna la vita sociale di ciascuno di noi, i ragazzi possono stare a scuola e non devono più stare a casa, con gli enormi problemi che, anche dal punto di vista

Credo che votando contro il Governo, com'è accaduto stamani, probabilmente non lo saremo, ma non lo dirà la prossima tornata elettorale. A noi lo dirà qualcosa di ben più importante di un voto nei prossimi mesi o nel prossimo anno e mezzo, o quando sarà: se siamo stati all'altezza del dare un Paese sicuro da tutti i punti di vista alle prossime generazioni, ai nostri figli e ai nostri nipoti, lo diranno soltanto i fatti; non saranno le elezioni a dirci che abbiamo fatto bene, ma lo sapremo soltanto se i nostri figli e i nostri nipoti saranno sicuri prima di tutto dal punto di vista della salute e, poi, dal punto di vista economico; anzi, insieme dal punto di vista economico. Questa è una sfida. Il Partito Democratico sa dove stare, lo ha dimostrato in questi due anni e continuerà a dimostrarlo. Se ci venite dietro farete un piacere a tutto il Paese.

gentile sottosegretario Sileri, cari colleghi senatori, intervengo ancora una volta in dichiarazione di voto - ne sento tutta la responsabilità - su un decreto che va convertito

di quanto la strategia di contrasto alla pandemia da Covid-19, messa in atto dal Governo Draghi, ha avuto successo.

di sale da concerto, di locali di intrattenimento musicale ed altro ancora, in zona bianca addirittura al 100 per cento, lo si deve ad una campagna di vaccinazione che ha avuto successo. ha avuto successo. Il Governo ha inteso accogliere le richieste delle Regioni italiane e della Conferenza delle Regioni perché evidentemente il CTS, che supporta scientificamente il Governo Draghi, ha ritenuto che tali richieste oggi, o meglio quando è stato approvato il decreto capienze, potessero avere accoglienza e potessero essere approvate nel Governo Draghi e poi evidentemente consegnate al Parlamento, perché il decreto-legge venisse convertito nei termini previsti dalla nostra Costituzione. quindi, che questo sia un giorno particolare, al di là delle polemiche che sono nate nel corso della discussione per l'approvazione degli emendamenti, sui quali si è discusso e votato anche in 1a Commissione. Questo è un giorno positivo, perché è la dimostrazione che, così come ha correttamente e abilmente narrato nel suo intervento il collega Luigi Vitali, il Governo italiano si è saputo distinguere in efficacia e in efficienza rispetto al contrasto alla pandemia da Covid-19, facendo meglio di altri Paesi occidentali e di altri Paesi dell'Unione europea, che invece hanno agito che spesso in passato veniva attribuita al *modus operandi* degli italiani. Invece noi abbiamo dato dimostrazione di essere un Paese serio, che si affida a persone qualificate e competenti. Non dimentichiamoci - e lo voglio ricordare ancora una volta - che l'affidamento della responsabilità della campagna di vaccinazioni al generale Figliuolo è stato un grande successo ed è giusto ricordarlo, perché questa è stata la prima delle importanti scelte che hanno adottato Mario Draghi e il Governo che egli presiede. discorso vale, ovviamente, per la Protezione civile, che ha affiancato il generale Figliuolo in questa campagna, e per le Regioni che gli sono state dietro: bisogna fare un plauso alle Regioni per quanto hanno saputo fare e alle città, che hanno seguito un percorso

Poi vedremo se non l'hanno fatto per paura del vaccino o perché ideologicamente no vax e quindi e quindi collocati in quell'alveo di persone che pensano che, a prescindere da tutto, i vaccini facciano male sempre e non solo quello contro il

per il Governo di ottenere, in questa circostanza, il voto favorevole di una maggioranza parlamentare molto ampia, che evidentemente ha saputo apprezzare i successi di quanto accaduto in Italia in questi mesi,

e di grande rigore, come la Germania, l'Austria e l'Olanda, che invece oggi, purtroppo, proprio a causa di una bassa percentuale di vaccinati, la pandemia con provvedimenti di restrizione della libertà personale molto severi. Ciò evidentemente contrasta con un modo di fare solitamente molto più serio, che che in questo momento pone invece l'Italia ai vertici, come Paese guida, come Paese da prendere ad esempio, caro Sileri, per il senso di responsabilità degli italiani e di tutta l'organizzazione sanitaria.

*(Applausi)*. Adesso dispiace verificare come gli altri Paesi ci abbiano creduto un po' meno e ora stiano combattendo contro la quarta ondata. Purtroppo, anche in Italia, nonostante nonostante una percentuale molto alta di vaccinazioni, dobbiamo riscontrare un aumento dei contagi. Ieri, improvvisamente, i positivi sono schizzati ad oltre 10.000. Noi non possiamo, quindi, sottovalutare questo aspetto. Leggevo che gli esperti virologi sperano che il punto più alto della svolta di di questa nuova ondata di Covid-19 possa arrivare il prima possibile, per consentire agli italiani di vivere un Natale e delle festività natalizie in santa pace. È evidente, però, che dobbiamo essere molto attenti e solerti, capire che non possiamo permetterci di abbassare la guardia. È questa la ragione per la quale il Governo ha spesso detto no ad emendamenti che tendevano ad aprire ulteriormente, c'è anche un atteggiamento di prudenza. L'atteggiamento del Governo tiene conto, ovviamente, dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico. Noi dobbiamo credere nella scienza; dobbiamo credere nei medici. Sono troppi i colleghi, troppi i colleghi, anche qui in Senato, che vorrei si iscrivessero alla facoltà di medicina, perché hanno una propensione naturale a capire di medicina, quando, invece, hanno magari sì e no una laurea

degli esseri umani, soprattutto degli italiani, è cresciuta di circa venti anni negli ultimi cinquanta anni, voi capite bene che non è un caso. O ci crediamo o non ci crediamo. Quando ero bambino sono stato vaccinato;

Come dicevo l'altro giorno in Aula, io mi sono fatto somministrare la terza dose, perché erano trascorsi sei mesi dalla seconda, e l'ho fatto volentieri. Io sono qui ad affermare che tutte le polemiche, delle quali mi dispiace, messe messe in piedi da chi è intervenuto per dichiarazione di voto per il Partito Democratico, non hanno senso. I voti espressi su due emendamenti, con il parere contrario del Governo, non sono un segnale contro il Governo, cara sottosegretario Bini. Erano due questioni di merito. La prego di voler recepire quanto le sto dicendo: Forza Italia non ha votato contro il Governo. Ha votato a favore di due emendamenti.

che il nostro voto favorevole è un voto favorevole al Governo e che i voti sugli emendamenti nulla hanno a che vedere con il progetto di

Signor Presidente,forse è bene che il senatore Pagano stia anche a sentire, oltre che ricevere i complimenti del suo Gruppo.

di cercare di portare fuori il Paese dalla situazione di pandemia. Questo è uno dei decreti-legge con cui si danno delle indicazioni, anche importanti, per la ripresa

questo senso di responsabilità, in cui ognuno ha le sue idee - perché c'è sempre il merito - in cui ognuno presenta i propri emendamenti e delle opzioni, avendo una visione diversa, ci siamo confrontati. Il problema però è che non può

è proprio il Ministro di Forza Italia che dice di no e poi il Gruppo Forza Italia con grande gioia vota contro il parere del Governo. mi dovete spiegare come si sta in questa maggioranza. Sappiamo tutti che ognuno di noi fa parte di questa maggioranza solo per la situazione del Paese, perché la pensiamo in maniera diversa e abbiamo valori diversi.

che tutti insieme, collettivamente, ci dobbiamo far carico della situazione. Colleghi, stiamo scherzando col fuoco. Non siamo in una situazione tranquilla. Qui sono tutti tranquilli, ma non dovete stare tranquilli, perché i contagi stanno riprendendo e c'è una situazione che dobbiamo attenzionare. Ancora non ne siamo fuori e,

capire esattamente qual è il principio di responsabilità nei confronti del Paese e serve capire fino in fondo come si sta in questa maggioranza, perché non ci possono essere alcuni che devono sempre farsi carico di tutto, subire e magari votare cose che non condividono e altri che interpretano liberamente il loro ruolo di parlamentari. Siccome però qui siamo tutti parlamentari e abbiamo le nostre idee, se questa è la linea, ognuno la interpreterà

Presidente, colleghi, il Senato è chiamato oggi a esaminare e convertire il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139. È chiaro a tutti che ci troviamo in presenza di un provvedimento dal forte impatto sociale e che rappresenta un altro sostanziale passo verso quella normalità che come Lega auspichiamo e caldeggiamo ormai da molti mesi, normalità perché, tra le tante e troppe privazioni e ferite che in questi mesi di pandemia ci hanno inferto, la più profonda e lacerante è probabilmente proprio la perdita della nostra normalità, dei piccoli gesti, delle nostre consuetudini. Abbiamo pungolato il Governo e il Parlamento giorno dopo giorno, provvedimento dopo provvedimento, proprio per raggiungere risultati importanti per il nostro Paese e per chi aspetta risposte da noi. In questi mesi abbiamo raccolto migliaia di istanze che ci arrivavano da imprenditori, commercianti, lavoratori, pensionati, studenti o semplici cittadini in difficoltà e abbiamo provato a dar loro voce con tutte le nostre forze. Siamo orgogliosi di essere riusciti a muovere alcuni passi nella loro direzione, pur essendo consci che il lavoro da fare è ancora molto. Il decreto che oggi quest'Assemblea è chiamato a esaminare apporta sostanziali modifiche in svariati settori e l'appellativo di decreto-legge capienze, come si è deciso di rinominarlo per una sorta di semplificazione lessicale, non ritengo possa rappresentare appieno la vera portata del provvedimento. Nel testo infatti sono previste, non solo importanti novità sul fronte delle riaperture, ma anche norme sulla riorganizzazione e sul rafforzamento della pubblica amministrazione, norme in materia di esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, norme per l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia e disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Sinceramente in materia di capienze, pur ribadendo che il tema della sicurezza deve essere sempre quello predominante, avremmo auspicato una maggiore uniformità di azione. Non possiamo fare a meno, infatti, di notare e rimarcare alcune incongruenze che continuano a lasciarci perplessi. Giusto per citare un esempio ben rappresentativo del concetto, penso all'emendamento presentato dalla collega Pergreffi e da altri colleghi, che chiedeva per i bus turistici una capienza completa limitata ai soggetti possessori del certificato verde, proposta poi accolta dall'Assemblea, ma che non era stata accettata dal Governo con motivazioni che fatichiamo a comprendere, considerato che per aerei e treni a lunga percorrenza è già prevista questa possibilità, mentre per il trasporto pubblico locale non è nemmeno richiesta la certificazione verde. Registriamo favorevolmente la decisione dell'Assemblea di accogliere anche il nostro emendamento che prevede di vincolare alle necessità del solo popolo afghano le risorse aggiuntive per il fondo di asilo previste dal decreto. Come Gruppo siamo assolutamente sensibili alle difficoltà che stanno vivendo migliaia di donne, uomini e bambini afghani e ritenevamo importante scongiurare ogni possibilità che i fondi previsti potessero poi venire utilizzati per finalità differenti da quelle originariamente previste, facendo venir meno l'aiuto del quale il popolo afghano ha assoluta necessità. Se un decreto-legge interviene per attivare 3.000 posti nel sistema di accoglienza in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, è perché si riscontrano la necessità e l'urgenza di far fronte alle esigenze dei profughi afghani, che il nostro Paese ha accolto e sta accogliendo tramite canali ufficiali. allora non specificarlo in modo chiaro nel testo, all'insegna del buonsenso e della trasparenza, così da evitare che le risorse aggiuntive possano essere direzionate altrove? Esprimo altresì soddisfazione per l'accoglimento del nostro ordine del giorno teso a contribuire e a ridare slancio a un settore - quello dell'attività fieristica - che è stato uno dei più colpiti dalla pandemia e che rappresenta un comparto fondamentale per l'economia del nostro Paese. Una menzione a parte merita, per le importanti e impattanti novità proposte, l'articolo che ritengo maggiormente complesso e, se vogliamo, interessante per il suo contenuto, cioè l'articolo 9, contenente disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Signor Presidente, non nascondo che l'originaria stesura dell'articolo 9 ha sollevato parecchi dubbi e perplessità, considerato l'impatto delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali, che necessitavano di una limitazione dello scopo perché non indirizzate solo a casi specifici o alle missioni per il PNRR, riferentesi alle comunicazioni di dati tra soggetti pubblici senza previa autorizzazione del Garante e senza ulteriori basi normative di legge o di regolamento. Queste e altre criticità sono state sottolineate nelle diverse audizioni svolte in Commissione affari costituzionali, che hanno sollecitato un intervento necessario rispetto all'originaria formulazione dell'articolo. Desidero congratularmi pubblicamente con il relatore del provvedimento, collega Augussori, per il lavoro di sintesi e sinergia che è riuscito a portare avanti su un tema così delicato, proponendo, di concerto con il Governo e gli altri organi interessati, una riscrittura dell'articolo 9 che ci sembra più equilibrata e che è la perfetta risultanza di un lavoro svolto con totale professionalità. Credo che questo possa essere considerato un esempio di come il Parlamento, sfruttando appieno tutte le sue capacità, debba e possa ancora ricoprire il ruolo centrale ed essenziale che gli spetta e che deve sempre pretendere di ricoprire. In tal senso, esprimo soddisfazione per l'accoglimento di un nostro emendamento volto a rendere effettiva la tutela dell'utente telefonico attraverso l'utilizzo del registro delle opposizioni, destinato a raccogliere le richieste di tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse e mobili. Con tale modifica si completa l'assetto sistematico delineato dall'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, rendendo operativo lo strumento della revoca del consenso eventualmente prestato anche per le chiamate automatiche. Il tema della *privacy* dei nostri cittadini è per noi della Lega primario e imprescindibile ed è per questo che siamo attenti a ogni dettaglio. Sappiamo infatti che su temi così delicati non sono ammissibili fraintendimenti o leggerezze. È proprio in tale ottica che desidero focalizzare l'attenzione sulla modalità di trattamento dei dati sanitari e sulla profilazione che, se non effettuata correttamente, potrebbe portare a una disapplicazione di fatto della normativa vigente. La profilazione è una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati riservati consistente nell'utilizzo degli stessi per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione e gli spostamenti. quindi dire che l'attività di profilazione si compone di un trattamento automatizzato che ha uno svolgimento su dati personali e finalità valutativa degli aspetti personali di una persona fisica. È facile comprendere la natura invasiva di quest'attività, che può comportare danni e abusi a carico degli utenti se il titolare del trattamento dati non adotta particolari cautele, a maggior ragione se si parla di dati sanitari...

L'obiettivo di questa operazione è certamente nobile e condivisibile. Si punta infatti a costruire nei prossimi anni un moderno sistema sanitario in Rete tra tutti i soggetti cittadini, in grado di modificare concretamente il funzionamento della sanità pubblica e migliorare l'importante azione della prevenzione attiva, incidendo anche sull'economicità della spesa. Non dobbiamo però dimenticare che un simile trattamento deve avvenire sempre per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante nell'ambito della sanità pubblica e che in ogni caso l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto solo a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) che produca effetti giuridici che lo riguardano e che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona. In conclusione, anche se avremmo preferito che una tale tematica fosse stata trattata in un apposito provvedimento,

Si tratta di una legge molto importante e delicata che deve, da una parte, permettere il rilancio del sistema produttivo del nostro Paese dopo i gravi danni subiti a causa del blocco delle varie attività dovuto alla pandemia dall'altra, deve tenere conto del contesto sanitario che stiamo vivendo che non ci permette ancora, purtroppo, di poter abbassare la guardia. L'approccio del MoVimento 5 Stelle verso le misure legate alla pandemia da Covid-19 è sempre stato improntato al massimo di precauzione rispetto alla situazione epidemiologica. Fin dal principio con la guida del Governo Conte II abbiamo costruito un sistema fondato sulla responsabilità, sulla collaborazione sistematica con la comunità scientifica e sulla proporzione delle misure rispetto alla situazione sanitaria. Oggi, per fortuna, ci troviamo in uno scenario diverso. Purtroppo, non possiamo dire di aver sconfitto il nemico Covid-19, ma vediamo bene la luce fuori dal *tunnel*. Grazie alla campagna vaccinale iniziata quasi un anno fa, grazie a comportamenti responsabili da parte dei cittadini e grazie ai progressi dei protocolli di cura abbiamo recuperato in parte la normalità della nostra vita quotidiana. Non dobbiamo disperdere questo formidabile patrimonio di strutture, filiera sanitaria, conoscenze e comportamenti virtuosi, ma siamo anche in una fase in cui, mai come oggi, ogni misura adottata e ogni decreto-legge approvato deve essere improntato a criteri di equilibrio, proporzionalità e adeguatezza. Interventi sproporzionati in senso restrittivo suscitano la comprensibile rabbia di cittadini e imprese che vengono da quasi due anni di sacrifici incalcolabili. «Le misure vanno dosate con equilibrio, se introduci una misura sovradimensionata c'è una reazione del Paese. Se non sono misure percepite come necessarie e adeguate, la popolazione non ti viene dietro». Sono le parole che il nostro presidente Giuseppe Conte ha pronunciato all'assemblea di Confesercenti e che condivido. Conte ha aggiunto: «Il *green pass* credo sia una buona soluzione, oggi ci consente di affrontare questa quarta ondata con la dovuta sicurezza» ma «sono contrario a operare ulteriori strette». Teniamo ben presenti queste parole perché ci permettono di mantenerci ragionevoli in una situazione ancora complicata. Come detto, il provvedimento affronta molteplici temi che sono stati esaminati nel corso dell'esame presso la 1a Commissione, che ha migliorato che ha migliorato le disposizioni presenti. Grazie, in particolare, al lavoro del Movimento sono state approvate diverse misure importanti, in primo luogo quella che apporta una modifica alla legge di bilancio 2017 al fine di escludere dall'obbligo di utilizzo del biglietto nominativo le manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati e rievocazioni storiche o similari, le giostre per accesso a spettacoli e strutture con una capienza superiore a 5.000 spettatori. Si tutela, quindi, un settore importante per il nostro Paese che era in evidente situazione di svantaggio. Sul tema dello svolgimento delle fiere in presenza in zona bianca e gialla, come dei convegni dei congressi e la loro relativa capienza, è stato accolto un nostro ordine del giorno e speriamo che presto il Governo possa tenere fede all'impegno. altro argomento abbiamo molto discusso in Commissione. Mi riferisco all'articolo 9, che reca disposizioni in tema di *privacy* e tutela dei dati. In merito ad esso molte associazioni hanno a cuore questa tematica; si sono esposte e hanno dibattuto sulla carta stampata e sui *blog* evidenziando come l'argomento sia fortemente seguito e sentito. La norma originaria introduceva uno sproporzionato ampliamento delle condizioni che legittimano il trattamento dei dati personali, necessario all'esercizio di poteri pubblici o nell'interesse pubblico. Infatti, si prevedeva che le pubbliche amministrazioni potessero definire autonomamente le basi giuridiche e le finalità del trattamento dei dati personali se connesse all'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge capienze, invece, il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni era consentito solo se vi era un espressa norma di legge che lo autorizzava. È bene evidenziare che il Garante della *privacy* nei suoi interventi ha ribadito la necessità di una norma di rango primario che autorizzasse il trattamento dei dati personali dei cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni, proprio invocando la previsione dell'articolo 2-*ter* del codice *privacy* per i trattamenti che presentano rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, quelli previsti dall'articolo 2-*quinquiesdecies* che conferivano al Garante un potere di intervento preventivo al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini. L'abrogazione di tale potere di intervento, accompagnato all'ampliamento dei poteri della pubblica amministrazione, secondo la prima formulazione della norma, creava aree di rischio per i diritti e le libertà dei cittadini ove le valutazioni effettuate dal Garante negli interventi preventivi non venissero attuate internamente alle pubbliche amministrazioni. Detto ciò, la *ratio* della novella è chiara: consentire uno snellimento rispetto alle condizioni che legittimano la pubblica amministrazione a effettuare trattamenti dei dati personali nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali, uno snellimento senz'altro auspicabile in ragione dell'importante mole di progetti che inevitabilmente le pubbliche amministrazioni sono chiamate a gestire in questo particolare periodo, ma che si consuma al di là della contingenza come cambiamento di sistema, destinato a incidere permanentemente sulla disciplina vigente. Se l'esigenza di una semplificazione è senz'altro condivisibile, l'emergenza sanitaria non può, però, travolgere qualsiasi baluardo di protezione dei diritti dei cittadini, come nel caso in questione. Per rimediare a tali distorsioni, come Gruppo MoVimento 5 Stelle siamo intervenuti con una serie di emendamenti che sono stati recepiti dal relatore e dal Governo, che hanno riscritto l'articolo 9 del provvedimento. *(Applausi)*. Sulla base delle nostre proposte, in primo luogo, anziché eliminare la necessità di base giuridica per il trattamento, è stato ampliato l'elenco delle possibili basi giuridiche, aggiungendo gli atti amministrativi generali. Un simile intervento non comporta un appesantimento degli oneri dei soggetti pubblici eventuali titolari dei trattamenti, giacché impone loro semplicemente l'adozione di un atto amministrativo di portata generale, attraverso il quale identificare le caratteristiche del trattamento che si ritiene necessario intraprendere per il perseguimento delle finalità istituzionali loro attribuite dalla legge. Inoltre, è stato recuperato il ruolo del Garante anche nella fase di *post* approvazione: si prevede - ad esempio - che, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva - e comunque nei casi di adozione di decreti-legge - il Garante esprima il parere in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge oppure in sede di esame definitivo degli schemi di decreti legislativi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari. Con i nostri subemendamenti abbiamo definito meglio la norma, allungando da nove a dodici mesi i termini entro i quali i gestori delle piattaforme digitali conservano il materiale oggetto della segnalazione in tema di *revenge porn* soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Infine, abbiamo sostenuto il potenziamento del ruolo organico con relativo stanziamento di risorse per l'Autorità garante. Come sancito anche quest'anno dal *digital economy and society index* (DESI), l'Italia si conferma ancora all'ultimo posto in Europa per competenze digitali avanzate. Ed è anche a causa di questo che rimane - a mio parere - la persistenza di un pregiudizio che attanaglia le pubbliche amministrazioni e il settore produttivo del Paese, ossia che la norma sulla *privacy* sia un ostacolo alla semplificazione e alla trasformazione digitale, un onere burocratico e amministrativo da eliminare. Spesso, invece, la normativa risulta male interpretata. Il fine è consentire l'uso del trattamento di dati per innumerevoli fini leciti, ma allo stesso tempo di eseguire tali trattamenti in modo corretto, considerando sempre prioritariamente il dovere etico di tutelare i diritti delle persone coinvolte. In conclusione, colleghe e colleghi, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e mi auguro che questo provvedimento venga presto convertito in legge.

che riesce a mettere dentro pezzi di riorganizzazione del Ministero della salute; temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e quant'altro. Insomma, ci sono tante norme che dentro il decreto-legge capienze fanno fatica a essere inserite e, quindi, mi sembra proprio una spinta. Oggi, per la prima volta abbiamo avuto un sussulto di dignità da parte del Parlamento, che si riappropria del suo ruolo centrale, umiliato e frustrato costantemente dal voto di fiducia che il povero ministro D'Incà è costretto a porre

abbiamo provato a rimetterci un po' al centro e a far capire al Governo che, anche se si cerca in nome dell'emergenza di tenere tutti buoni, fuori c'è un Paese che ha bisogno di risposte. Qualche rispostina in più abbiamo tentato di dare: ecco perché abbiamo votato favorevolmente su alcuni emendamenti. Nel suo impianto, però, questo decreto-legge è fuori sincrono rispetto al Paese e alle esigenze degli italiani. Ho sentito dire ancora una volta la storia: «Vi abbiamo riconosciuto la libertà di vaccinarvi o meno». Poi, però, se ci avvaliamo di quella libertà, ecco che abbiamo un prezzo da pagare. Se viene riconosciuta la libertà e il diritto anche a non avvalersi della vaccinazione, non capisco il motivo per cui mi vogliate o ci vogliate togliere anche un solo milligrammo di tale libertà. Questo è il tema politico di fondo e credo che avremo ancora modo e tempo di parlare di tutti i limiti che ci imporrete. Ringrazio quindi il Parlamento e i colleghi, perché per la prima volta abbiamo dato dimostrazione di

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri è stata celebrata la Giornata mondiale della prematurità e del bambino nato prematuro. Monumenti e ospedali illuminati di viola, video, convegni e tavole rotonde che riuniscono professionisti del settore e rappresentanti dei genitori genitori sono alcune delle iniziative organizzate dalla Società italiana di neonatologia per promuovere e attenzionare le complesse problematiche, ma anche i grandi passi avanti fatti dalle terapie intensive neonatali del nostro Servizio sanitario nazionale, i quali permettono oggi quasi dei miracoli. Le nuove tecniche di rianimazione cardiopolmonare e un'assistenza sempre più accurata permettono oggi di salvare anche neonati estremamente pretermine. Sono più di 30.000 i nati prematuri solo nel nostro Paese ogni anno. ieri abbiamo celebrato la grande forza e la voglia di vivere di questi piccoli combattenti e delle loro famiglie. È un segnale importante, diamo voce alle famiglie dei piccoli pazienti, che ogni giorno vivono e convivono con le tante problematiche con cui i loro piccoli eroi, i loro grandi amori, si trovano e si troveranno comunque a combattere in conseguenza della loro prematurità e delle complicanze a breve e lungo termine che talvolta residuano. Lo *slogan* «*zero separation*» vuole sensibilizzare sulla necessità di sostenere la vicinanza dei genitori ai loro neonati. I genitori non sono visitatori, ma parte integrante della cura. Con il coinvolgimento precoce della famiglia si rafforzano i legami e le connessioni emotive fondamentali per lo sviluppo neurocognitivo del bambino, i cui effetti positivi si potranno vedere a distanza. Contatto pelle a pelle e allattamento al seno rappresentano solo alcuni dei momenti essenziali per un migliore sviluppo del neonato in generale, ma in particolare di questi neonati. Tutto ciò deve sempre avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli anti-Covid. *Zero separation*, cioè la vicinanza genitori-neonato, va sostenuta e promossa: è incoraggiata da tutte le società scientifiche e dalla Società italiana di neonatologia *in primis*. Un grazie doveroso va a tutto il personale sanitario e parasanitario delle terapie intensive neonatali, che ogni giorno opera con sacrificio, competenza e professionalità per assistere questi piccoli esseri indifesi. Il 17 novembre è la giornata per un inno alla vita che nasce. *(Applausi)*.

È qualcosa che stiamo portando avanti da tempo, che per noi è importantissimo e rappresenta uno degli anelli fondamentali, se vogliamo effettuare una vera transizione. Tra ritardi e rinvii burocratici, l'Italia non è ancora al passo nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica, nonostante la legge di bilancio per il 2021 imponesse di realizzare una rete di infrastrutture di ricarica ad alto potenziale entro il 30 giugno 2021, ma allo stato attuale il piano di realizzazione è bloccato. Considerato che la transizione energetica poggia su due pilastri fondamentali (le politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto circolante e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sia sulla rete stradale sia sulle autostrade), senza questi strumenti sarà difficile raggiungere gli obiettivi europei e soprattutto sarà molto difficile effettuare una transizione nel settore dell'*automotive*.

all'ordine del giorno. Dalle notizie che stanno trapelando pare ci sia un aumento del contagio. Noi, attraverso questa interrogazione, chiedevamo esattamente la anche per incentivare il vaccino, evitando gli obblighi surrettizi e l'inasprimento dei toni legati al *green pass*, su cui dovremmo fare una riflessione.

ricoverati in terapia intensiva e, purtroppo, deceduti tra coloro che erano vaccinati e coloro che non lo erano. Soprattutto adesso che si è dato il via alla terza dose, addirittura anche sugli *over* 40,

Mi sento di chiedere al Ministro alcune cose. La prima: perché non ha ancora risposto? La mia quindi è una speranza,

la sensibilità che il Ministro dimostra nei confronti di quel Paese. in questi giorni abbiamo appreso dalla stampa che il ministro Cartabia ha chiesto al suo omologo statunitense di far tornare in Italia Chico Forti. Una nota diffusa dal Ministero di via Arenula ha rinnovato la sua richiesta di trasferimento, affinché possa scontare nel suo Paese la pena cui è stato condannato in Florida, alla fine di un processo per omicidio dai contorni nebulosi, ricco di falle e privo di prove concrete a suo carico. Ringrazio di cuore il ministro Cartabia per il suo lavoro e mi auguro che continui a tenere alta l'attenzione su questo caso drammatico, per far sì che possa avere almeno un lieto fine. Signor Ministro, le chiedo di andare avanti con tenacia. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo senza perdere altro tempo. Era infatti il 23 dicembre 2020 quando il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio annunciava in modo plateale che Chico Forti sarebbe rientrato in Italia, forse sottovalutando la complessità della procedura. Il 29 marzo successivo, lo stesso Ministro faceva sapere che Forti sarebbe stato trasferito in un altro penitenziario, al quale verrebbero assegnati detenuti in attesa di trasferimento. Da allora non abbiamo saputo più nulla, nonostante il nostro Paese aspetti con ansia il rientro di Chico Forti e la sua famiglia combatta da oltre vent'anni contro quello che sembra un enorme errore giudiziario, che ha letteralmente distrutto la vita sua e di tutti quelli che gli vogliono bene. Il 16 giugno scorso, signor Presidente, ho presentato un'interrogazione per sapere cosa sarà di Chico. Nessuno mi ha risposto. Oggi, a distanza di un anno dall'annuncio in pompa magna fatto dal ministro Di Maio, rinnovo la mia richiesta al Governo di avere risposte, ma qui in Aula e non a mezzo stampa. Quindi, signor Presidente, tramite lei chiedo al Governo, al ministro Cartabia e allo stesso ministro Di Maio di venire a rispondermi. Non lo devono fare per me, ma per Chico Forti, per la sua famiglia sua famiglia e per tutti quelli che si sono affezionati a lui, pur non conoscendolo, e che vogliono aggiornamenti sulla sua triste vicenda. Nell'attesa di ricevere una risposta, infine, voglio fare un appello al presidente Draghi, consapevole della stima di cui gode a livello internazionale e dell'onestà intellettuale che lo contraddistingue. Presidente Draghi, faccia qualcosa. Aiuti Chico Forti a ritornare nel suo Paese. Nessuno potrà mai risarcirlo; la sua famiglia non potrà essere neanche risarcita per gli anni che le sono stati rubati e per tutto il dolore che ha vissuto. Se c'è stata però un'ingiustizia, in qualche modo va sanata. Presidente Draghi, intervenga. Chico da oltre vent'anni aspetta che il nostro Paese gli tenda una mano.

Presidente, voglio portare alla vostra attenzione due casi emblematici sul mancato riequilibrio dei divari che ancora attanagliano il nostro Paese. Ricordo che il riequilibrio dei *gap* territoriali è uno degli obiettivi indicati espressamente dall'Unione europea e che quindi siamo tenuti a rispettarlo. Il primo caso riguarda proprio le fondazioni bancarie. Ci risulta che la Compagnia di San Paolo, di origine torinese, abbia progettato una Next generation We a beneficio esclusivo di alcuni municipi, quelli del Nord-Ovest: una sorta di sistema di supporto nei servizi per aggiudicarsi i bandi del PNRR. Voglio far notare che l'istituto creditizio controllato dalla Compagnia di San Paolo, che peraltro è Intesa San Paolo, che ha rilevato rilevato anche il Banco di Napoli, opera in tutta Italia e all'estero ed è molto presente nel meridione, anche grazie alle vecchie filiali anche del Banco di Napoli. Come funziona, allora, il risparmio in Italia? I conti correnti dei meridionali vanno bene, ma, quando si tratta di ridistribuire le risorse, si pensa solo ad alcuni Comuni, quelli di casa propria. Ricordo tra l'altro che, su 86 fondazioni presenti in Italia, solo dieci si trovano al Sud, svantaggiato pure nella capacità di attrazione dei fondi, come se non bastasse tutto il resto. L'andazzo però non riguarda solo la Compagnia di San Paolo: anche altre fondazioni si stanno regolando così; basti vedere cosa accade con Monte dei paschi di Siena. Passiamo al secondo caso, che riguarda il fondo per l'abbattimento delle liste d'attesa inserito nel disegno di legge di bilancio di previsione. Ci risulta che la Regione che ne beneficerà più di tutti sarà proprio la Lombardia, in generale il Nord, e che al Sud andrà solo il 33,4 per cento, secondo i calcoli. Ora, se questa divisione con il bilancino può sembrare a prima vista corretta, nei fatti non lo è. È risaputo che a soffrire maggiormente per le liste d'attesa siano proprio le Regioni del Sud, tanto è vero che i cittadini meridionali sono spesso costretti a veri e propri viaggi della speranza per curarsi:

Signor Presidente, a nome di tutti i cittadini del Sud, chiedo quindi conto pubblicamente, sia al Governo, sia al Parlamento, di questi due fatti, che giudico gravissimi e che ci dicono che la strada per l'uguaglianza è ancora molto lunga. **Atti